Onorevoli colleghi, come già preannunciato ai Gruppi per le vie brevi, comunico che venerdì 17 dicembre alle ore 11,30 il Ministro dell'interno renderà un'informativa all'Assemblea sugli incidenti avvenuti a Roma nella giornata di martedì 14 dicembre.

novembre 2010, n. 187, è stato esaminato in prima lettura dalla Camera dei deputati che ha modificato il testo introducendo alcune disposizioni. legge di conversione è stato votato in Assemblea con l'astensione dei Gruppi di opposizione e senza nessun voto contrario, a dimostrazione di una generale convergenza sugli obiettivi del provvedimento, al di là di ogni possibile contrapposizione politica. D'altra parte, i temi affrontati riguardano questioni e problematiche di straordinario rilievo: la sicurezza dei cittadini, la lotta alla criminalità organizzata...

la sicurezza dei cittadini e la lotta alla criminalità organizzata rappresentano sfide decisive per lo Stato. Ad esse siamo chiamati tutti a concorrere, in uno sforzo comune che possa produrre frutti duraturi. Presso le Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia il testo non ha subito modificazioni. Riferisco quindi brevemente sui contenuti del decreto-legge, nonché sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, poi svolgere anche alcune considerazioni sull'intesa raggiunta tra i Gruppi parlamentari circa la discussione e l'esame di alcune importanti questioni sulle quali erano stati assunti impegni formali in Parlamento già in sede di approvazione del piano straordinario antimafia. Il capo I del decreto reca misure per gli impianti sportivi, in particolare con riferimento ai reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, nonché in relazione agli obblighi in capo alle società sportive di garantire la sicurezza nei propri stadi, anche con l'uso di personale *ad hoc* (i cosiddetti *steward*). Il capo II (dall'articolo 3 all'articolo 5) reca disposizioni per il potenziamento dell'attività di contrasto alla criminalità organizzata e della cooperazione internazionale di polizia. In particolare, l'articolo 3 introduce misure volte al sostegno dell'attività dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati. Ricordo che il comma 3 prevede che l'Agenzia possa essere autorizzata dal Ministro dell'interno a stipulare contratti di lavoro a tempo a tempo determinato, in deroga alla dotazione organica prevista dalla sua legge istitutiva. A seguito di una modifica apportata dalla Camera dei deputati, l'Agenzia potrà altresì avvalersi di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle agenzie (compresa l'Agenzia del demanio) e dagli enti territoriali, assegnati all'Agenzia medesima anche in posizione di comando o di distacco. Avendo ritirato, al pari di tutti i colleghi, i miei emendamenti, ho presentato due ordini del giorno: con il primo si chiede al Governo di assicurare che il personale distaccato presso l'Agenzia sia adibito in ogni caso a mansioni equivalenti a quelle svolte presso l'amministrazione di provenienza. Con il secondo si impegna parimenti il Governo a garantire

previste dalla normativa vigente, ossia l'evidenza pubblica e non le chiamate a titolo personale. L'articolo 5 istituisce il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia. Il capo III reca invece disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare norme di interpretazione autentica di alcune disposizioni del piano straordinario antimafia che, su alcuni particolari aspetti, viene anche puntualmente integrato con norme volte, tra l'altro, a rendere più incisiva ed efficace la normativa sulla tracciabilità. Il Capo IV si occupa della sicurezza urbana. Il Capo V detta, infine, disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno. Come preannunciato, adesso desidero ora svolgere alcune considerazioni circa il possibile percorso comune che è stato individuato nella seduta svolta questa mattina presso le Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia. I senatori dei Gruppi di opposizione, fin dall'inizio dell'esame in sede referente del provvedimento, avevano posto all'attenzione della maggioranza e del Governo una questione di particolare rilievo, connessa all'impegno assunto dall'Esecutivo durante l'esame in Senato del cosiddetto piano straordinario antimafia. In quella occasione, nella seduta del 3 agosto scorso, era stato approvato un ordine giorno, senatori Vizzini, Bianco, Berselli, Della Monica, D'Alia, Li Gotti, Bodega e Pistorio (espressione quindi di tutti i Gruppi parlamentari), con il quale il Governo si impegnava, tra l'altro, a sostenere la discussione e l'approvazione di una serie di di legge in materia di reati di associazione di stampo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, autoriciclaggio e scambio elettorale-politico mafioso, nonché misure sui collaboratori di giustizia ed altri interventi volti a rendere più rapido ed efficace il procedimento di adozione delle misure di prevenzione patrimoniale. Il decreto-legge attualmente al nostro esame è stato discusso in prima lettura dalla Camera dei deputati senza che nessuna di queste materie sia stata introdotta in quella sede. Nel momento

che ha stabilito che anche per gli emendamenti ai decreti-legge sono necessari i requisiti di necessità e urgenza, e anche perché formali richiami sono venuti di recente anche da parte del Presidente della Repubblica

sottolineare che la questione posta in quegli emendamenti era seria: una questione nella quale non si può non riconoscere una ragione nel merito da parte dei colleghi che li hanno presentati. Su questo argomento si è discusso a lungo nella mattinata di oggi. Voglio ringraziare per il contributo dato al nostro dibattito il Ministro dell'interno,

che rappresentavano le stesse istanze che io ho cercato di rappresentare. Si è pensato che una soluzione avrebbe potuto essere quella che i Gruppi ritirassero tutti i rispettivi emendamenti al decreto-legge

velocità nell'esame del disegno di legge per arrivare entro la prima settimana di febbraio all'approvazione del provvedimento in questo ramo del Parlamento per poi trasmetterlo all'altro ramo. Su questa soluzione si è trovata un'intesa ragionevole che ci consente oggi di affrontare le questioni sul tappeto dando una risposta pronta, così come pronta è stata quella della Camera dei deputati che ha approvato il provvedimento senza voti contrari, ma non vanificando lo sforzo che insieme dobbiamo fare per affrontare problemi che sono altrettanto urgenti e che, pur senza lo strumento della decretazione d'urgenza, saranno affrontati in tempi brevissimi, mi auguro (come sempre in questa materia) con l'impegno di tutti i Gruppi parlamentari.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, intervengo come Presidente della Commissione giustizia del Senato per quanto riguarda le questioni di nostra competenza. Il decreto-legge in conversione rappresenta un ulteriore passo lungo la strada del ripristino della sicurezza pubblica, intrapresa fin dall'inizio della legislatura con una serie di provvedimenti, tra i quali si segnalano, in particolare, il decreto-legge n. 92 del 23 maggio 2008, convertito dalla legge n. 125 del 24 luglio dello stesso anno, recante misure urgenti in misura di sicurezza pubblica; il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori; la legge 15 luglio 2009, n. 94, il cosiddetto pacchetto sicurezza; il decreto-legge n. 4 del 4 febbraio di quest'anno, convertito dalla legge n. 50 del 31 marzo, che ha istituito l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; infine, il piano straordinario contro le mafie e la delega al Governo in materia di normativa antimafia, approvati con la legge 13 agosto 2010, n. 136. Per quanto riguarda le disposizioni di più diretta competenza della Commissione giustizia da me presieduta, il comma 3 dell'articolo 2 dispone l'applicabilità ai reati di violenza o minaccia nei confronti degli dell'aggravante prevista dall'articolo 339, terzo comma, del codice penale, di fatto commesso «mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone». Il comma 4 equipara gli *steward* ai pubblici ufficiali, al fine dell'applicazione delle pene previste per il reato di lesioni personali gravi o gravissime ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive (in particolar modo l'articolo 583-*quater* del codice penale). La Camera ha precisato che l'applicazione della disposizione si riferisce all'espletamento delle mansioni svolte dagli *steward* in occasione delle manifestazioni sportive. Si segnalano anche le disposizioni per il potenziamento dell'attività di contrasto alla criminalità organizzata e della cooperazione internazionale di polizia di cui al capo II, ed in particolare l'articolo 3, che introduce misure volte al sostegno dell'attività dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati, e l'articolo 4 che integra la commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di protezione e vigilanza con un magistrato designato dal Ministro della giustizia, tutte le volte in cui la commissione sia tenuta ad esprimersi su questioni di sicurezza relative a magistrati. Opportunamente, la Camera dei deputati ha specificato che il magistrato che va ad integrare la composizione della commissione deve essere designato fra quelli già collocati con incarico fuori ruolo presso il Ministero della giustizia. Dopo un proficuo e aperto confronto nelle Commissioni 1a e 2a riunite, con la fondamentale e decisiva presenza del ministro Roberto Maroni, si è giunti ad una totale condivisione del contenuto di una legge di conversione, approvata - come ha giustamente ricordato il presidente Vizzini - senza voti contrari dall'altro ramo del Parlamento. Si è convenuto in particolare, su proposta sempre del presidente Vizzini, di affrontare urgentemente - ripeto: urgentemente - in altra sede le questioni ancora aperte, e su ciò vi è stato l'impegno esplicito della maggioranza e anche e soprattutto del ministro Maroni.

All'unanimità il Senato ha accolto questa posizione, allora del Partito Democratico, e l'invito del ministro Maroni a

pubblici; la questione relativa alle squadre investigative comuni internazionali; quella relativa al riciclaggio e all'autoriciclaggio, una materia importante e delicata che concerne anche l'ordinamento della polizia locale, quindi una serie di misure destinate anche in quell'ottica; infine, la questione dell'autodenuncia per quanto riguarda i reati di usura. Ebbene, oggi abbiamo accettato questo impegno, pronunciato all'interno delle due Commissioni e poi anche oggetto di comunicato stampa da parte del ministro Maroni,

e dal collega Casson il percorso che è stato fatto e l'impegno del ministro Maroni su questo tema, che non è nuovo, anche nel concordare alcune questioni che ci stanno fortemente

più volte è stato anche in quest'Aula detto e noi stessi abbiamo plaudito al successo che le forze dell'ordine e la magistratura hanno portato in tanti campi (penso alle azioni contro la criminalità organizzata, ad alcuni eccellenti arresti, all'assicurazione alla giustizia di tanti latitanti) di dire che personalmente non mi convince l'impianto complessivo non di questo provvedimento, bensì di come noi stiamo affrontando in questo Paese i temi della sicurezza e tutte le questioni ad esso connesse. Non mi convince perché, ancora una volta, di là della condivisione delle singole norme così come in questo provvedimento, noi ci troviamo sempre ad affrontare provvedimenti che contengono tante norme messe insieme in campi molto disparati. Penso - come in questo caso - alla sicurezza negli stadi, al Fondo di solidarietà civile, all'Agenzia per i beni confiscati, alla tracciabilità dei flussi finanziari, alle gestioni commissariali e alle disposizioni sugli enti locali. Insomma, signor Ministro, le chiedo e mi chiedo: sarebbe stato possibile affrontare in un provvedimento organico tutto il tema, per esempio, dell'Agenzia per i beni confiscati? Sarebbe stato possibile affrontare il tema della tracciabilità dei flussi finanziari in modo organico? Sarebbe stato possibile affrontare il tema della sicurezza urbana senza che questa si disperdesse in tanti e tanti provvedimenti ai quali abbiamo assistito? Io credo di sì. Si potrebbe discutere sulla qualità della legislazione che produciamo, ma credo anche del disordine normativo che talvolta deve correggere se stesso, come anche in questo caso in alcune parti del provvedimento, e del carattere episodico e talvolta anche propagandistico di molte norme. Certo alcune disposizioni sono state migliorate, in questo come in altri provvedimenti, nei passaggi tra Camera e Senato e anche nel merito sono state da noi condivise, dunque, come per esempio in questo caso, il nostro voto di astensione alla Camera è stato così motivato. Pur tuttavia, intendo soffermarmi su un punto di critica politica relativamente, come ho detto in precedenza, a un impianto ahimè emergenziale che ha caratterizzato gli interventi in tema di sicurezza. A questo si aggiunge una critica di merito, perché spesso le questioni della sicurezza non sono state poi una priorità in termini di risorse economiche, di riorganizzazione e di riassetto delle forze dell'ordine impegnate nel contrasto alla criminalità. Preciso inoltre che molte norme, che appunto da noi sono state anche condivise (e molte altre potevano essere migliorate), portano sicuramente il segno della nostra proposta, ma l'intero impianto sicuramente non è sistematico e dobbiamo rispondere talvolta a questo problema, altre volte ad un altro problema emergenziale, perdendo la visione d'insieme. Gli interventi che il Governo ha proposto nel corso del tempo non hanno previsto quindi, a mio avviso, un intero assetto normativo di idea, di pensiero, di cultura politica sui temi della sicurezza, oltre - ripeto e voglio sottolinearlo - alle risorse poco credibili e spendibili, operando invece continuamente tagli che hanno minato la credibilità e la possibilità di attuare azioni di contrasto capillare e diffuso sui territori. Nonostante queste difficoltà siamo grati, l'ho detto anche all'inizio del mio intervento, alle forze dell'ordine, alla magistratura, ai successi ottenuti in questo campo. Tutto ciò non è sufficiente e non può bastare: la sicurezza, quella dei nostri territori, quella di tutti i giorni necessita di un'azione costante, capillare, non solo di operazioni eccellenti; necessita di mezzi, di risorse, di nuove e più qualificate professionalità. Purtroppo in questo campo non abbiamo riscontrato grandi interventi, non solo per i richiamati tagli del Governo, ma anche per le difficoltà quotidiane che si debbono affrontare in termini organizzativi. Eppure, signor Ministro, è da quando è stata varata la riforma costituzionale che, nello spirito e nella lettera della nostra Costituzione, si pone all'ordine del giorno la necessità e credo anche il dovere per i legislatori e per il Governo di affrontare il tema di una legge nazionale di coordinamento tra le competenze tra i vari livelli istituzionali, in particolare per raccordare con una legge ordinaria i poteri e le competenze che discendono dal nuovo assetto costituzionale (penso agli articoli 117 e 118). Non si tratta solo di una questione giuridica e di assetto e di struttura dell'impianto normativo, quanto di una più profonda esigenza di tipo culturale, politico e istituzionale, quella cioè di mettere finalmente in campo una visione e un intervento normativo che delinei un sistema integrato, e in particolare mi riferisco alla sicurezza urbana. Il Ministro lo sa e sa che da molti anni questo tema viene affrontato in Europa e in Italia da molti operatori, da molti enti locali e da molte Regioni, ma finora è mancato un intervento governativo e del legislatore di vero coordinamento e di integrazione tra sistemi e risorse per poter dare luogo ad azioni efficaci e significative per tessere quella rete di azioni necessarie a rendere più visibile ed esigibile la sicurezza urbana nelle nostre città. In molti anni e in altre sedi ci siamo anche incontrati sul versante della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome o dell'ANCI sulla necessità di organizzare un sistema integrato di sicurezza e molte proposte avanzate in quelle sedi oggi giacciono in Parlamento noi ci auguriamo che vengano esaminate al più presto. Infatti, vede, signor Ministro, stiamo producendo una miriade di azioni che però, a mio avviso, non hanno una visione d'insieme; inoltre, il continuo proliferare di questi interventi potrebbe portare al sovrapporsi di poteri e di strumenti, mancando il coordinamento e rischiando addirittura di creare confusione. L'esempio più lampante è costituito dalla scarsa valenza e dalla non condivisibile idea - almeno a mio avviso - delle ronde; un'idea non solo poco attuabile, ma che avrebbe invece potuto trovare risposte molto più serie in una visione improntata all'allargamento e al concorso alla sicurezza urbana anche in termini di sicurezza partecipata,

e poi abbandonata dai Governi successivi, soprattutto da quelli di centrodestra, che invece avrebbero dovuto prevedere un monitoraggio delle azioni effettuate loro messa a sistema, attraverso una legislazione di coordinamento nazionale che facesse dialogare i vari livelli istituzionali in modo coerente. Ma in questo Paese spesso si perde traccia delle cose positive e si ricomincia sempre da capo, forse anche e solo perché si rappresenta un altro schieramento politico, ed è molto difficile consolidare un tessuto comune su alcuni punti fondamentali. Un ulteriore esempio potrebbe essere rappresentato dalla scorciatoia dei poteri che abbiamo attribuito ai sindaci con le ordinanze: poteri che gli stessi sindaci hanno richiesto, sicuramente perché verso di loro si indirizzano pressioni e domande urgenti sui territori e si pretendono risposte. Però anche in quel caso, signor Ministro, si poteva ragionare in termini di sistema ed evitare di volta in volta il sovrapporsi di poteri in mancanza di risorse per i Comuni, con tagli alle azioni di prevenzione. Faccio un esempio per tutti: le mancate risorse in termini di prevenzione nel campo dei minori con il Ministero della giustizia ulteriori fondi per il controllo degli spazi pubblici. Molti altri esempi potrebbero essere portati al fine di avvalorare quello che ho detto in questa sede. Mi preme sottolineare come tante azioni, talvolta anche qualificate, rischiano di disperdersi se non sono tenute insieme da una visione integrata di un nuovo sistema di sicurezza

i propri ruoli, ma non ciascuno per sé e ognuno da solo come avviene oggi. Signor Ministro, in conclusione credo che il salto di qualità ci obbligherebbe ad un ragionamento molto più complesso, ad un riordino di tanti comparti, a partire da quelli enunciati in questo stesso provvedimento; pertanto, pur condividendo molte norme, la sua estemporaneità e la mancata capacità di esprimere norme di riordino omogenee e complessive mi rende difficile condividerne la *ratio* ispiratrice e l'impianto che lo permea.

il concerto di maggioranza e opposizione, con il parere positivo del Governo, lo scorso agosto. Allora si aveva ancora la speranza che nel giro di qualche mese, cioè entro il 30 novembre, come è scritto nell'ordine del giorno, si sarebbe passati

che, tranquillizzati gli animi, ha caratterizzato il dibattito delle Commissioni riunite 1a e 2a di questa mattina troverà qualche ostacolo nelle prossime settimane. Infatti, se dopo gli impegni solenni assunti nell'agosto scorso dal Ministro ci dovessimo trovare a fronteggiare un decreto-legge che tratta vari argomenti - probabilmente necessari, anche se sicuramente non urgenti - credo che ci sarebbe di che stare attenti sia in sede di Comitato ristretto che successivamente, quando si passerà alla rassegna dei disegni di legge e si avvierà un lavoro di preparazione del testo unico.

sul conferimento di ulteriori poteri agli *steward*, una sorta di legione straniera che verrà armata (fortunatamente non dal punto di vista della dotazione bellica)

all'interno di un contesto come quello di una partita di qualsiasi livello, ci sarà di che divertirsi nelle prossime settimane, nel momento in cui questo decreto-legge diventerà legge, visto e considerato che all'interno degli stadi ancora si può parlare. Sappiamo che non si possono più manifestare le proprie idee per iscritto, ma oralmente è ancora possibile farlo, è possibile urlare. Siamo in un contesto in cui, negli ultimi 15 anni, sono state adottate misure sempre più restrittive della libertà personale all'interno di una manifestazione sportiva, conferendo poteri incontrollabili

Abbiamo ritirato gli emendamenti, e questo è un fatto. Non si capisce fino a quando andremo avanti con il dibattito e quando eventualmente verranno posti all'attenzione dell'Aula altri documenti, come per esempio alcuni ordini del giorno presentati in Commissione, che mi sono permesso in parte di ripresentare anche in Aula,

circa l'accesso alle manifestazioni sportive stesse. Ad oggi, infatti, tutto quel che avviene nell'applicazione di quell'articolo va contro la Costituzione. Si chiede anche di raccomandare ai prefetti l'emanazione di ordinanze che non discriminino sulla base, di sesso, età e provenienza geografica, l'accesso alle manifestazioni sportive. È successo più volte, nelle settimane scorse, che i non residenti non potessero andare a vedere la partita, con la conseguenza ricordata anche dal presidente Vizzini in Commissione. Infatti, non avendo questa fantomatica tessera del tifoso si è costretti ad andare in un settore che non è quello destinato alle squadre ospiti, mettendo così tifoserie rivali nello stesso settore. Chiedo infine di di modificare l'articolo 9 della legge n. 41 del 2007, prevedendo una scadenza temporale della data del divieto di accesso nei casi sopra descritti. Tutto ciò viene promosso

Signor Presidente, le relazioni che abbiamo ascoltato sono sicuramente esaurienti

che, nell'arco di due anni, per cinque volte si intervenga con misure urgenti significa che ci si muove spesso a macchia di leopardo, senza una visione organica della materia; mentre alcuni temi, che pure sono condivisi, in fondo sono stati nel tempo accantonati. Oggi, in Commissione,

incidenti nell'ambito di manifestazioni sportive: quindi l'urgenza è motivata), abbiamo deciso di ritirare i nostri emendamenti, che non erano altro

da una quota (pari ad un quinto) del Fondo unico giustizia di pertinenza del Ministero dell'interno.

cento del totale; sicché, al Fondo unico giustizia, affluisce 100, al Ministero dell'interno 10.

Questo Fondo di solidarietà civile va a gravare per la misura di un quinto della quota del Fondo unico giustizia di pertinenza del Ministero dell'interno: ossia, ossia, la quota di pertinenza del Ministero dell'interno si riduce all'8 per cento. Quel fondo doveva servire a potenziare i servizi, la quotidianità del lavoro delle forze dell'ordine: non solo, invece, è stato defalcato nel corso delle diverse leggi, sino alla legge n. 2 del 2009, che ha rappresentato un taglio notevole, ma ora questa risorsa viene ulteriormente defalcata, perché un ulteriormente defalcata, perché un quinto deve andare al Fondo di solidarietà civile. Questa è una norma che noi vogliamo modificare, perché riteniamo che il Fondo unico giustizia debba essere ripartito tra il Ministero essendo il risultato dell'attività della magistratura e delle forze dell'ordine, essendo il risultato, il prodotto in termini economici, del lavoro

o sequestrati - perché sono beni che producono utili - si dice che quegli utili che affluiscono al Fondo unico giustizia vengono assegnati

la gestione di risorse che sono estremamente necessarie alla funzione istituzionale del Ministero della giustizia. Per il resto, non posso che ribadire la fiducia nell'impegno assunto dal Governo e dai Presidenti di Commissione, sperando di poter, in tempi brevi, arrivare all'introduzione nel nostro ordinamento di quelle norme

lavoro (approfitto per stigmatizzare il fatto che pochi Ministri seguano da vicino i nostri lavori). È suo preciso dovere, soprattutto nella misura in cui si viene a chiedere una cortesia istituzionale come in questo caso. Sempre come considerazione preliminare, vorrei insistere con una richiesta che ho già fatto in Commissione, perché alla fine di questo nostro dibattito lei ci dia un'informativa sui fatti di ieri.

che questa Aula si accontenti della ricostruzione che lei già ha: se non è completa, venerdì ci fornirà la doverosa appendice. Infatti, essere qui, cari colleghi, a discutere un provvedimento sulla sicurezza, sicurezza, prevalentemente negli stadi, senza avere nemmeno una sommaria informativa del Ministro dell'interno su quello che è successo ieri in questa città, città, nel cuore di Roma, fatti che sono sulle prime pagine di tutti i giornali, mi sembra una cosa difficilmente comprensibile. La prego di non rispondermi in termini formali dicendo che ha bisogno delle 48 ore. l'opinione pubblica si sta formando sulle notizie che circolano. Sarebbe bene che, seppur in termini cautelari, una parola del Ministro nella sede istituzionale più alta, che è la nostra, incominciasse a ricostruire i fatti, se non a dare un giudizio politico. Per tornare al nostro provvedimento, voglio solo riprendere alcuni dei temi che sono già stati molto ben individuati e messi alla nostra attenzione, in particolare, dalla collega Incostante. Ci troviamo ancora una volta a discutere di un decreto-legge da convertire con scadenza incombente, che reca nel titolo: «misure urgenti in materia di sicurezza». In realtà, come i colleghi hanno ascoltato dai nostri nostri due relatori, il provvedimento parla di sicurezza negli impianti sportivi, di potenziamento dell'attività di contrasto alla criminalità organizzata e della cooperazione internazionale

Continuare a predisporre tanti decreti d'urgenza sulla sicurezza vuol dire che non abbiamo un quadro organico dei problemi e che non stiamo mettendo mano a nessun vero e forte progetto di riforma.

di chiederle per quale ragione i nostri emendamenti, che trattavamo esattamente delle questioni i cui titoli ho prima richiamato, siano inaccoglibili, mentre l'insieme del decreto-legge è ai sensi della nostra Costituzione, cioè avrebbe i requisiti di necessità e urgenza. È un ragionamento onestamente

Nel merito delle questioni, vorrei solamente soffermarmi su un punto, che ritengo abbastanza esemplificativo del fatto che non possiamo continuare a procedere in questo modo e che abbiamo bisogno di una riforma organica del comparto, in applicazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, come ben diceva la senatrice

della Repubblica: e se andate avanti così finalmente si ricostituirà anche l'unità di CGIL CISL e UIL (l'aspetto). Un'unità così delle sigle sindacali delle forze dell'ordine non si era mai vista quella dei Corpi: dai Vigili del fuoco alla Polizia, con i Carabinieri che non potendo fare le manifestazioni mandano però i loro messaggi

come anticipato dai colleghi che mi hanno preceduto, contiene degli spunti positivi. Ma, a mio parere, occorrerebbero elementi correttivi su alcune questioni importanti che sono strumentali al contrasto della criminalità: sull'Agenzia per i beni confiscati, per esempio, e sulle misure che attengono alla tracciabilità dei flusso finanziari. In particolare, per quanto riguarda l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati occorrerebbero correttivi per farla funzionare al meglio e potenziarla. In particolare, sarebbe opportuno che nei Comuni con meno di 15.000 abitanti i beni sequestrati e confiscati potessero potessero essere destinati direttamente in concessione per finalità sociali agli organismi privati che assicurano la maggiore garanzia per il perseguimento dell'interesse pubblico. In questo modo si risolverebbe una delle maggiori difficoltà incontrate dall'Agenzia, e cioè la presenza di beni sequestrati e confiscati che non riescono ad essere assegnati perché nei piccoli Comuni, dove spesso c'è un forte inquinamento dove spesso c'è un forte inquinamento della criminalità organizzata, i sindaci sono sovente soggetti a pressioni che non consentono loro di procedere all'assegnazione dei beni.

stessa si autofinanzi anche con la gestione dei patrimoni aziendali confiscati o sequestrati alla mafia. Questo forse è uno degli aspetti più importanti della realtà economica delle organizzazioni criminali e rappresenterebbe, da un lato, una via di finanziamento importante, dall'altro, un modo per conoscere la gestione contabile delle aziende che sono proprie del patrimonio delle organizzazioni criminali, oltre che un modo per dare visibilità e utilità all'azione dello Stato e un messaggio certo alle organizzazioni che gestiscono le imprese economiche che andrebbero a finanziare proprio l'Agenzia nata per la lotta contro la criminalità. Altro punto focale importante riguarda la tracciabilità dei flussi finanziari. Questo meccanismo è stato messo a punto nella legge n. 136 del 2010, votata anch'essa all'unanimità dal Parlamento, che ha visto un'attività di costruzione operosa nell'ambito della Commissione di riferimento, cioè la Commissione giustizia. Essa prevede una delega al Governo per l'emanazione di un codice delle misure di prevenzione nei confronti della mafia, ma pone anche norme immediatamente precettive riguardanti proprio la tracciabilità dei flussi finanziari. Per quanto concerne la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, pure condivisibile, voglio sottolineare l'opportunità di un suo rafforzamento attraverso l'introduzione di una norma per far assumere gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi anche ai subappaltatori e ai subcontraenti, subcontraenti, a pena di nullità dei contratti. La tracciabilità dei flussi finanziari per gli appalti può e deve diventare uno strumento efficace di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni criminali nel tessuto economico legale (soprattutto in questa fase di crisi economica) e deve essere affiancata da nuovi interventi legislativi, come ad esempio l'introduzione del reato di autoriciclaggio del denaro proveniente da attività criminali e misure contro il voto di scambio. In particolare, la previsione dell'autoriciclaggio come reato appare una riforma necessaria se si vuole operare un efficace contrasto alla criminalità organizzata. Sarebbe sufficiente prevedere che il patto di scambio può essere rappresentato da un'altra un'altra utilità, oltre che dal denaro. Infatti, la condotta di riciclaggio da parte dell'autore di un altro reato, grazie al quale ha incamerato profitti illeciti, deve essere un'altra condotta punibile: se si rimediano soldi con manovre oscure e, poi, senza trasferirli a terzi, li si reinveste in prima persona, dovrebbe essere naturale essere puniti per tale condotta. Punire il reato di autoriciclaggio è dunque una necessità assoluta. desidero ricordare che siamo l'unico Paese in Europa a non prevedere come reato il reinvestimento di capitale illecitamente percepito da parte dell'autore del primo illecito: si tratta di uno strumento essenziale per la lotta alle mafie, che nel nostro ordinamento ancora oggi non esiste.

*(PdL)*. Signor Presidente, il decreto-legge che è arrivato oggi in quest'Aula, dopo essere stato approvato lo scorso 2 dicembre alla Camera è di fondamentale importanza per diversi aspetti della sicurezza nel nostro Paese, in quanto sono tante le questioni che abbraccia, e tutte molto rilevanti. Anzitutto, parlando di sicurezza, non possiamo che rendere merito al ministro dell'interno, onorevole Maroni, per il lavoro che sta facendo da quando ha ottenuto l'incarico e per la lotta alla criminalità, grazie alla quale, tra le altre cose, questo Governo si è distinto alla guida del Paese. Viviamo in tempi di grande allarme sociale. I terribili scontri di ieri a Roma dimostrano che l'asticella si è alzata e sempre più facinorosi sono pronti a dare l'assalto alle nostre istituzioni, al nostro Parlamento e alla nostra libertà. È mia opinione che in questo caso lo Stato di diritto debba manifestare tutta la forza che gli dà la legge, per far sì che i colpevoli delle devastazioni nel centro di quella che è una delle città più belle del mondo e patrimonio della cultura italiana vengano portati di fronte alla giustizia e scontino le pene che devono scontare. I giornali e le televisioni hanno riportato la notizia che tra i *black block* e gli pseudomanifestanti c'erano anche degli infiltrati di alcuni gruppi ultras, e non certo infiltrati della polizia, come peraltro è stato detto. Abbiamo visto di recente quanto è successo a Genova a settembre durante l'incontro tra l'Italia e la Serbia, a che punto la follia e la violenza di questi individui possono arrivare. Il Governo e il Ministero dell'interno sono visti come nemici da questi gruppi di criminali: essi vedono in noi uno strumento di limitazione dei loro poteri, che in passato sono stati anche più grandi di adesso, a causa delle politiche *soft* dei Governi precedenti e della contiguità tra alcuni partiti e i più estremisti dei gruppi ultras. Quest'oggi tutto ciò non esiste più. Il Governo ha deciso di occuparsi della questione del tifo violento già con alcuni strumenti utili per filtrare gli ingressi negli stadi: dai tornelli alla tessera del tifoso, aspramente combattuta proprio perché limitativa del potere di questi scalmanati. Ora, con il decreto che arriva oggi in Aula, aggiungiamo altri due tasselli nella lotta contro la violenza negli stadi: l'arresto in flagranza di reato e l'equiparazione degli *steward* a pubblici ufficiali negli stadi. Troppo spesso abbiamo visto in passato le nostre valorose forze dell'ordine assaltate, proprio come è successo ieri a Roma e a Genova, durante Italia-Serbia, da gruppi di teppisti disinteressati allo sport e da gente che va allo stadio solo per creare disordini. Il nostro intento non è solamente repressivo, anzi. Con questo decreto-legge si cerca di portare una cultura della sicurezza nei nostri impianti sportivi che prevenga le violenze e non solo le reprima. Gli stadi, gli impianti sportivi devono essere luoghi in cui le famiglie e la gente comune va per divertirsi, per svagarsi, per passare una domenica all'aperto. Non si può essere ostaggi di personaggi che sono liberi di scorrazzare a loro piacimento perché nessuno li può punire. Tutto ciò non è più tollerabile per una società civile, democratica ed aperta. Vi è poi il capitolo relativo all'immigrazione, secondo quanto richiesto dalla Commissione europea per rendere più omogenea la normativa relativa alla lotta alla clandestinità. Solo grazie ad un coordinamento tra tutte le Nazioni europee ci si può opporre ad un vero e proprio mercato di uomini, che non si può certo combattere con la demagogia o un malinteso buonismo. Di ciò va dato atto al Governo che ha sempre svolto una politica incisiva su questo tema, aprendo all'immigrazione con criterio e dando spazio a chi vuole entrare in Italia per lavorare e non per delinquere. Rilevante, anche considerando la crisi finanziaria che ha colpito l'Occidente, è la norma relativa alla rintracciabilità dei pagamenti, mezzo fondamentale per andare a scoprire chi, dietro l'uso di una carta plastificata, perpetra truffe ai danni della società e di tutti noi. Un altro provvedimento su cui il Ministro si è impegnato anche oggi nelle Commissioni affari costituzionali e giustizia è quello relativo al pacchetto autoriciclaggio, ai rapporti tra politica e criminalità, al cosiddetto voto di scambio e, infine, al rapporto tra lo Stato e i collaboratori di giustizia. Si tratta di materie molto complesse che troveranno il loro spazio in discussioni più ampie, che coinvolgeranno sicuramente anche l'opposizione in un rapporto di reciproca collaborazione. deputati questo provvedimento ha ottenuto un'ampia maggioranza. Le forze politiche hanno espresso un grande senso di responsabilità mostrando che la politica, quando serve, sa anche decidere con celerità sulle questioni che più stanno a cuore ai cittadini. Siccome quest'Aula si è sempre distinta per il suo alto profilo istituzionale, sono convinta che sapremo discutere e votare questo decreto-legge prima che la decadenza renda inutile questo percorso.

assiste ad un primo segno di responsabilità generale. Un dato importante è che tutti i Gruppi parlamentari hanno unanimemente deciso di varare il più velocemente possibile questo provvedimento,

in sede amministrativa dal Ministero. Vorrei ricordare il grande sforzo che abbiamo sostenuto per licenziare le norme sul contrasto all'immigrazione clandestina, le modifiche apportate ai nostri codici per l'introduzione del reato di immigrazione clandestina, che ha consentito una maggiore efficacia nel reprimere

l'inasprimento di tutte le pene per le violenze effettuate nei confronti dei soggetti che chiamiamo deboli, donne. Infine, vi rammento il grande potere offerto in materia di sicurezza urbana a tutti i nostri sindaci. A questo punto, basta che usino detto strumento eccezionale dell'ordinanza onnicomprensiva,

Far funzionare al meglio l'Agenzia per l'amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata è un fatto basilare, rappresenta la chiusura del cerchio. Ricordiamo che

semmai quei soggetti hanno usato la mafia per vendere qualche libro in più e per fare affari, accusando altri di non fare ciò che devono fare.

controllo di tutti i flussi finanziari, dai pagamenti agli incassi. Ebbene, noi crediamo che sia questo il vero fenomeno da combattere, quello che più preoccupa e danneggia l'economia sana del nostro Paese.

indurre a pensare che, inevitabilmente, il nostro Paese sarebbe stato un Paese con una demografia d'immigrazione perennemente

colleghi: li possiamo leggere come vogliamo, ma sono dati! E tutto sommato l'immigrazione complessiva è calata del 40 per cento. Credo che questi dati li abbiamo letti tutti, perché non sono di anni fa, ma di ieri. Per questo, signor ministro Maroni, noi non possiamo che ringraziarla e invitarla a continuare su questa strada. Buon lavoro. finestra") *(PD)*. Signor Presidente, signor Ministro, in due anni e mezzo il Governo ha presentato tre decreti-legge e un disegno di legge in materia di sicurezza. Un numero così elevato di interventi in materia dimostra che è necessario predisporre un provvedimento legislativo organico, se si vuole superare una gestione emergenziale dei problemi. Il decreto-legge si occupa di quattro temi principali: la sicurezza urbana, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la tracciabilità dei flussi finanziari e la sicurezza delle manifestazioni sportive. Alla Camera dei deputati il Partito Democratico, dichiarando il proprio voto di astensione, ha tenuto a sottolineare che, malgrado le modifiche apportate al testo e quindi alcuni miglioramenti, non era possibile prescindere dalle caratteristiche del provvedimento definite da una forma e da un contenuto. La forma è il ricorso allo strumento del decreto-legge, mentre il contenuto è costituito dalla sostanza del decreto-legge n. 187 che, pur contemplando alcune norme condivisibili e più volte auspicate dal Partito Democratico, come quelle tese a dare operatività all'Agenzia dei beni confiscati e alla materia della tracciabilità dei flussi finanziari per il contrasto alla criminalità mafiosa contenuta nel Piano nazionale antimafia, presenta alcuni limiti. Li elenco. Innanzitutto, la questione della sicurezza viene affrontata con una logica emergenziale e non organica, senza dare risposte, ormai indifferibili, sia in relazione alle risorse per la sicurezza, sia per definire - alla luce della legge n. 121 del 1981 e degli articoli 117 e 118 della Costituzione - un sistema integrato di sicurezza che coinvolga, senza mortificarne la dignità, soggetti istituzionali a livello nazionale e locale con funzioni differenziate. In secondo luogo, vi è un'estensione di misure penali agli *steward*, che non è accompagnata da una definizione per legge ma piuttosto da un decreto del Ministro dell'interno dei nuovi compiti: non si comprende quali, ma certo non di polizia giudiziaria e non di pubblici ufficiali; nuovi compiti da assegnare quindi a soggetti che devono contribuire ad un servizio, ma certamente non ad un servizio pubblico. In terzo luogo, il tema dell'Agenzia dei beni confiscati è certamente affrontato, ma in termini che non ne garantiscono l'effettiva e da noi auspicata operatività e che destano perplessità sistematiche, venendo ancora una volta attribuita una funzione salvifica al Fondo unico giustizia, senza cogliere l'occasione di disporne per legge una ragionevole divisione tra giustizia e interno, in modo che ciascuno di questi comparti possa trarne risorse per autofinanziarsi. quarto luogo, il decreto affronta correttamente il problema della tracciabilità dei flussi finanziari, stabilendo che la normativa si applichi anche ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 136 del 13 agosto 2010. Tuttavia, l'originaria formulazione della normativa contenuta nel decreto, voluta dal Ministro dell'interno, ma anche dal Partito Democratico assolutamente condivisa, rischia di essere indebolita da alcuni emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati. Cito ad esempio l'introduzione di equipollenza di strumenti d'incasso, l'innalzamento dei limiti dei pagamenti in contanti da 500 a 1.500 euro, la previsione di un regime transitorio senza un termine finale condizionato all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e delle Poste, periodo durante il quale l'inserimento del CUP diviene facoltativo e non più obbligatorio. Ebbene, la tracciabilità dei flussi finanziari per gli appalti deve diventare, senza tentennamenti, uno strumento efficace di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni criminali nel tessuto economico-legale, soprattutto in questa fase di crisi economica. Il pacchetto di norme sulla tracciabilità è stato da noi ritenuto l'elemento qualificante del cosiddetto piano straordinario contro la mafia; per questo, avevamo presentato degli emendamenti, che abbiamo ritirato ma che speriamo possano essere recepiti in un altro atto legislativo. Ma questo pacchetto - è noto - avrebbe dovuto essere affiancato da altri istituti di contrasto alla mafia. Mi riferisco in particolare agli istituti inseriti nell'ordine del giorno G1, approvato dal Governo nella seduta del 3 agosto 2010, in cui divenne legge il cosiddetto Piano nazionale antimafia e su cui il ministro Maroni assunse fin da quella seduta un formale impegno di attuazione. Il Partito Democratico ritiene che sia importante che le norme incriminatrici del riciclaggio e dell'impiego di denaro, o beni o utilità di provenienza illecita, comprendano tra i soggetti attivi di entrambi i delitti in questione il concorrente nei reati presupposti, diversamente, non si consente l'incriminazione del cosiddetto autoriciclaggio, e questa esclusione suscita perplessità, sia a livello istituzionale, come capacità di contrasto all'economia illegale, sia nel contesto internazionale, con un'evidente necessità, tra l'altro, di adeguare di adeguare il sistema penale alle previsioni contenute nella terza direttiva europea antiriciclaggio. Inoltre, nel sistema vigente la nuova figura di reato di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall'articolo 416-*ter* del codice penale, circoscrive all'erogazione di denaro la controprestazione di chi ottiene la promessa di voti da parte della mafia con vantaggi a quest'ultima; ma la realtà criminologica dimostra che solitamente il politico cosiddetto appoggiato ricambia le organizzazioni mafiose con la concessione di favori differenti dal denaro. Analogamente, la disciplina dei collaboratori di giustizia ha trovato limiti nell'esperienza attuativa per la particolare rilevanza e complessità di talune collaborazioni, la pluralità degli impegni processuali a cui costoro sono chiamati, specie nella fase di avvio della collaborazione medesima. Occorre anche in questo caso intervenire e subito. Il Governo può e deve dare in questo campo, ed è estremamente importante per un salto di qualità nel contrasto alla mafia, un contributo anche nella ricerca di verità sulle stragi. Per questo avremmo voluto che Governo e maggioranza approvassero subito le modifiche indispensabili che avevamo proposto con i nostri emendamenti. Avremmo potuto farlo anche oggi, con un veloce passaggio alla Camera per una terza lettura e l'approvazione definitiva. Dobbiamo dimostrare alla mafia che vogliamo fare veramente un salto di qualità, quindi avremmo potuto farlo anche in quest'occasione. Su questi piani, come maggioranza e opposizione, possiamo e dobbiamo incontrarci. Abbiamo raccolto, signor Ministro, l'invito a ritirare anche oggi i nostri emendamenti. Sottoscrivendo l'ordine del giorno G1 il 3 agosto 2010, abbiamo ritenuto di fare un'apertura di credito nei confronti della maggioranza e del Governo, e lo abbiamo fatto anche oggi, perché siamo convinti che su una materia come questa il Parlamento non possa e non debba dividersi. Ci aspettiamo tuttavia che gli impegni che oggi lei, signor Ministro dell'interno, ha formalmente assunto nelle Commissioni riunite 1a e 2a, e che i presidenti Vizzini e Berselli hanno ricordato, vengano onorati entro il termine del 31 gennaio 2011, come da lei stesso suggerito.

che riguardava però gli interessi istituzionali del Paese e in cui il senatore Bianco è stato strettamente al mio fianco e deve essere sostenuto da tutti.

con cui la maggioranza ha affrontato il tema della sicurezza, che era stato declinato in campagna elettorale come un elemento fondamentale del programma di governo. In questi giorni si

è niente più che il compendio di una linea legislativa, di una politica del diritto con cui la maggioranza ha voluto riaffermare l'importante diritto alla sicurezza dei cittadini.

aveva illustrato più di 300 anni fa nel «Leviatano»: il fatto cioè che il diritto alla sicurezza rappresenta niente di più che il risvolto della medaglia dei diritti fondamentali di libertà. Con queste misure, signor Presidente, noi allarghiamo l'ombrello di protezione dei diritti fondamentali dei cittadini, interveniamo in materia di misure patrimoniali antimafia,

questa idea della sicurezza integrata rappresenta il culmine della politica del diritto e della sicurezza dei cittadini, perché in essa si dà attuazione a un principio costituzionale che che rinveniamo nell'articolo 114 della Costituzione, il cosiddetto principio del federalismo rafforzato o del regionalismo. cioè ai sindaci quegli strumenti attraverso cui le autonomie locali, in questo caso i Comuni, riescono a cooperare con le forze di polizia e lo Stato per realizzare questa idea della sicurezza integrata.

che in realtà si privava di un controllo democratico un potere che poteva incidere sui diritti fondamentali. Non è stato così: il controllo giurisdizionale operato dai giudici amministrativi ha dimostrato che solo in pochissimi casi, su 8300 Comuni, si era abusato di tale strumento. Con

di operare il coordinamento con le forze di polizia dello Stato. Le modifiche introdotte alla Camera prevedono che i Sindaci siano ufficiali di Governo e quindi rispondano del contesto e della struttura che la legge n. 121 del 1981 opera sul sistema di sicurezza dello Stato. Il Sindaco, quindi, ha il potere di emanare ordinanze in materia di sicurezza urbana; il prefetto, che ha un potere di ispezione sui sindaci, ha il potere di coordinare le forze di polizia dello Stato; il Ministro dell'interno, autorità nazionale di pubblica sicurezza, ha una funzione di coordinamento di tutte queste attività.

di quanto è stato fatto in Europa, in Francia, in Germania e nel Regno Unito, tra tutti i livelli istituzionali in cui si articola la nostra Costituzione. per un Paese democratico che ha fatto della sicurezza il rafforzamento dei presìdi di libertà, questo provvedimento non può trascurare neppure le altre misure in materia di antimafia, di cui non mi occupo perché porterebbe via molto tempo. È tuttavia necessario ricordare la realizzazione della banca dati del DNA ma soprattutto, nel disegno di legge collegato a questo decreto-legge, la possibilità di intervenire in materia di immigrazione clandestina comunitaria. Cercheremo di reinterpretare la direttiva comunitaria e intervenire in questi fenomeni, che conosciamo soprattutto sotto l'aspetto della prostituzione nelle strade urbane e del traffico di sostanze stupefacenti.

potremmo dimenticare che questo diritto alla sicurezza, e in questo caso la tutela dell'ordine pubblico, viene garantito da 450.000 operatori delle forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo dei vigili del fuoco, che da un po' di tempo rivendicano il riconoscimento della loro specificità. In questo provvedimento, signor Ministro, il Gruppo del Popolo della Libertà, a stragrande maggioranza dei suoi componenti, aveva presentato un emendamento finalizzato ad attribuire a detto personale il dovuto riconoscimento,

alla quantità e qualità del lavoro prestato, e al rischio, ed è oggettivo che questo personale rischi ogni giorno per difendere la libertà e la democrazia di questo Paese. Con questo il il Gruppo del Popolo della Libertà stigmatizza gli attacchi e l'azione politica violenta nei riguardi delle istituzioni, perché non sono trascorsi troppi anni da quando questi atti di violenza contro le forze dell'ordine si sono poi trasformati

Concludendo, ringrazio il relatore per questo importante provvedimento, e credo che dopo due anni e mezzo di legislatura, attraverso queste misure, abbiamo contenuto i livelli di criminalità, abbiamo allargato l'ombrello protettivo dei cittadini, abbiamo rafforzato le misure antimafia ed abbiamo arrestato un numero di latitanti che mai si era registrato nel nostro Paese. Cerchiamo di dare agli operatori delle forze di polizia e delle forze armate quel riconoscimento che mai era stato sottolineato in quest'Aula. Infine ricordo che, mentre noi cerchiamo di realizzare tali obiettivi, in quest'Aula era stata chiesta la creazione di commissioni di indagine sulle forze di polizia e la loro schedatura attraverso l'identificazione nelle uniformi. Il trattamento che noi riserviamo a questo personale è di grande rispetto e di grande dignità, perché credo che questo stia non nei codici di un partito politico, ma rientri nell'azione di governo. *(Applausi

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di

e che le risorse a copertura del comma 3 dell'articolo 3 siano riferite anche al personale comandato o distaccato presso l'Agenzia e non soltanto ai contratti a tempo determinato. Il parere è altresì dato nell'ulteriore presupposto che la norma di cui all'articolo 10 non comporti un aumento della spesa corrente per possibili promozioni, fermo restando il blocco dei *turn* *over* e di nuove assunzioni».

completo, ed aspettiamo gli Uffici, che l'hanno avuto all'ultimo momento. Però vorremmo essere in grado almeno di leggere gli ordini del giorno, per dovuta soddisfazione, per nostro dovere e nostro compito.

ad adottare le opportune iniziative al fine di garantire parità di trattamento agli appartenenti ai corrispondenti ruoli agenti, assistenti, sovrintendenti ed ispettori del Corpo della guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, che siano in possesso di tutti gli altri previsti requisiti per consentire la partecipazione al concorso pubblico per Commissario di pubblica sicurezza».

«a confermare le quote di attribuzione al Ministero della giustizia delle risorse». Dico questo perché com'è noto una decina di giorni fa il Consiglio dei ministri ha ripartito in

«impegna il Governo a valutare l'opportunità di provvedere», tenendo conto che già è stato fatto molto nella direzione prevista da questo ordine del giorno, sia dal Ministero della giustizia che dal Consiglio superiore della magistratura.

a indicare in modo preciso nel decreto ministeriale le mansioni di ausilio alle attività di polizia che gli *steward* saranno chiamati a svolgere».

il G102 è accolto

G115, senatore Perduca, c'è un invito al ritiro: accolgo l'invito. Si è sentito parlare molto di fiducia nel Governo. Chi ha fiducia nel Governo gli vota la fiducia; io ho votato la sfiducia a questo Governo e non mi fido delle parole pronunciate oggi in Commissione, tantomeno

complessivamente non lascia soddisfatti. Rispetto al quadro generale per noi rimane tutt'ora aperto, importante e fondamentale fondamentale il tema degli stipendi e delle dotazioni di mezzi per le forze dell'ordine, che da questo Governo continua a non avere risposte significative. Così come per noi rimane importante la non definizione e il mancato del Governo alla fase di regolamentazione del tema strategico della banca dati del DNA. Tuttavia, senza entrare nel merito degli aspetti del decreto che non ci convincono, ci teniamo a sottolineare, come abbiamo già detto durante la discussione alla Camera, gli aspetti positivi che il decreto pure contiene. In particolare, sottolineo il capitolo relativo alle norme antiriciclaggio, volte a contrastare le infiltrazioni mafiose nel settore degli appalti pubblici. Per questioni di residenza sono costretto a percorrere più volte

in cui non l'ultima impresa o l'ultimo cittadino, ma le migliori multinazionali e le imprese più importanti

con la criminalità organizzata, spesso utilizzando anche il sistema truccato del subappalto. Pertanto, l'introduzione dell'obbligo che costringe le ditte appaltatrici e subappaltanti ad indicare entro 180 giorni il codice unico di progetto per noi basterebbe per spingerci

l'intervento del collega Saltamartini un po' suscita l'esigenza

modo, nel momento in cui si parla di sicurezza, non possiamo dimenticare il malessere profondo che c'è nelle forze dell'ordine,

ha estratto la pistola pensando a chissà cosa succedeva. Noi dobbiamo manifestare la nostra solidarietà a chi difende la nostra sicurezza

l'UDC voterà a favore di questo provvedimento nella ferma convinzione che, quando si affrontano temi quali quello della sicurezza e della criminalità, debbano innanzitutto essere tenute in considerazione la gravità e la rilevanza del fenomeno. Occorre dunque cogliere queste occasioni come momento di coinvolgimento pieno di tutta l'Assemblea.

e vedere battersi il petto per i bellissimi - e nessuno più di me può congratularsi - arresti e sequestri, dimenticando che quelle norme sono state adottate da tutta l'Assemblea e che quegli arresti scaturiscono anche dall'attività dei magistrati e delle forze dell'ordine. Dispiace, quindi, non vedersi riconoscere questa collaborazione. Entrando maggiormente nel merito del provvedimento, ci appare condivisibile l'arresto in flagranza differita, così come l'impiego degli *steward*, misure in accordo con la consapevolezza che lo sport deve essere veicolo di valori positivi e non, come troppo spesso accade, occasione di violenza. Occorre un approccio chiaro e deciso nel trattare la gestione delle competizioni agonistiche negli stadi. Tuttavia, molto resta ancora da fare, in particolare sul fronte della prevenzione, ambito nel quale sarebbe utile garantire un maggior coinvolgimento delle società sportive e dei *club* e, mi consenta un piccolo suggerimento, evitare talvolta decisioni improvvide che finiscono per dare alibi ai violenti.

e di conseguenza, il divieto assoluto - e qua mi fa molto piacere perché sono contro questi divieti - ai tifosi della Roma di salire in quando si sa che tra tifoserie milanista e romane non corre buon sangue. Sono provvedimenti incomprensibili, talvolta, che danno alibi ai violenti. Attualmente i compiti degli *steward* sono individuati con un decreto del Ministro dell'interno del 2007 secondo cui le società di calcio devono impiegare per ciascuna gara un numero di *steward* non inferiore al rapporto di uno ogni 150 spettatori uno ogni 250 spettatori, in base alla capienza. La loro attività comprende, oltre alla bonifica dell'impianto, il prefiltraggio, il filtraggio e quant'altro. Il decreto oggi amplia tali compiti, anche se, a nostro avviso, in maniera troppo generica. Resta poco chiaro, infatti, quali possono essere gli ulteriori servizi ausiliari dell'attività di polizia relativa ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà. Per tale ragione, sarebbe indispensabile specificare, in futuri interventi legislativi, a quali servizi ausiliari ci si intenda riferire. Alcuni passaggi di questo provvedimento si sono resi necessari alla luce dell'approvazione del decreto del 2010 che ha istituito l'Agenzia nazionale per i beni sequestrati, e per la quale normativa - lo voglio ripetere - tutta l'Aula è stata partecipe e consenziente. Mediante tale istituto si sono volute colmare le attuali lacune, in direzione di un contrasto efficace ed efficiente alle mafie. Abbiamo apprezzato che il Governo abbia tentato di potenziare il personale nell'Agenzia, ma - a nostro avviso - esso non l'ha fatto in maniera adeguata. Il testo cita piuttosto vagamente la possibilità di avvalersi di personale in comando, in distacco o a tempo determinato. Appare prioritario garantire una professionalità e un canale di reclutamento adeguato, proprio in relazione alla delicatezza della materia. Allo stesso modo, ci lascia perplessi la possibilità di istituire ulteriori sedi dell'Agenzia. La scelta di Reggio Calabria non fu casuale, e una sede distaccata nella capitale era già prevista *ab origine*. Ma stentiamo a capire le ragioni di ulteriori duplicazioni. Le modalità di gestione dell'Agenzia devono caratterizzarsi per trasparenza, rendendo anzitutto pubbliche via Internet tutte le procedure di confisca e assegnazione dei beni. Altre perplessità sorgono in relazione alla norma che dispone l'integrazione della Commissione centrale consultiva per l'adozione di misure di sicurezza personale. In essa manca non soltanto un criterio di competenza del magistrato designato dal Ministro della giustizia, ma anche la previsione di una autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura. Analoghi dubbi emergono in riferimento all'istituzione di un nuovo Comitato per la cooperazione internazionale di polizia. Rafforziamo Rafforziamo gli uffici già esistenti - penso all'Interpol - estendendo i loro poteri, migliorando la loro funzionalità, nell'ottica di una sempre maggiore professionalità. Concordiamo appieno con le misure relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, che rappresenta uno degli strumenti più efficaci nel controllo degli appalti, per impedire in essi l'infiltrazione mafiosa. È altrettanto condivisibile, se non addirittura opportuna, la norma che prevede la predisposizione di una aliquota fissa di vice prefetti e vice prefetti aggiunti in posizione di disponibilità per i casi di conferimento di incarichi di gestione commissariale straordinaria, ovvero di incarichi connessi a specifiche esigenze di servizio o a situazioni d'emergenza. Essa può evitare che tali mansioni siano affidate a funzionari che abbiano altre incombenze. Con grande soddisfazione, infine, abbiamo preso atto della marcia indietro compiuta in relazione alla ambigua figura del sindaco sceriffo. L'articolo 8 del decreto-legge oggi in esame mostra con evidenza i limiti politici della scelta di attribuire ai sindaci poteri in materia di sicurezza. In quella sede, nel 2008, si sostenne il principio in base al quale la sicurezza dei cittadini possa derivare dalla scelta del sindaco quale ufficiale di Governo. Oggi ci si rende conto che la potestà sulle forze di polizia, senza le quali non si può discutere di sicurezza, non è concessa al sindaco, che deve necessariamente rapportarsi al prefetto. Concludendo, pur considerando il provvedimento non esaustivo, oggi esprimiamo - come già detto - una posizione favorevole. Si tratta di un sì che rappresenta una apertura di credito nei confronti di un Governo che si spera continuerà a lottare contro le mafie, così come fanno in silenzio tanti uomini e donne delle forze dell'ordine. Appena qualche giorno fa le proteste delle forze di polizia sono tornate a denunciare le gravi condizioni, signor Ministro, in cui versa

Manca il personale, non ci sono auto e si avverte la carenza di tecnologie e di formazione. Alcune caserme cadono persino a pezzi. Il comparto della Stradale è sotto organico per il 45

Ebbene, il nostro obiettivo è che la lotta alla criminalità organizzata non si traduca soltanto in dichiarazioni, ma si faccia costume e cultura, a partire da questo Parlamento, per coinvolgere l'intero Paese.

nei nostri territori. Allora, due anni e mezzo fa, non passava giorno che notizie riguardanti rapine, omicidi e stupri riempissero le pagine dei giornali. E di quel periodo, periodo, 2006-2008, ricordo i buffi tentativi del Governo Prodi nell'affrontare il problema della criminalità dilagante. In quel periodo tirava veramente una brutta aria. C'erano casi di omicidi efferati dal Nord al Sud dell'Italia.

Ho voluto citare solo i due casi più eclatanti. Sarà stato il triste provvedimento sull'indulto, che aveva fatto uscire dal carcere migliaia e migliaia di detenuti, saranno stati stati i cittadini extracomunitari clandestini che in parte, non trovando lavoro, venivano assoldati della criminalità, ma la verità è che quello è stato veramente un brutto periodo per la sicurezza dei cittadini nel nostro Paese. Oggi l'aria è cambiata. Oggi, dopo il duro e fruttuoso lavoro di questo Governo, in particolare del ministro Maroni, il Gruppo della Lega Nord è particolarmente soddisfatto dei risultati raggiunti nel campo della sicurezza e della lotta alla criminalità. Devo dire che non può che essere così: 18 miliardi di euro sequestrati e confiscati, quasi 7.000 arresti per reati di mafia, quasi tutti i 30 latitanti più pericolosi rinchiusi in carcere (gli ultimi due ancora in libertà, i famosi i famosi Matteo Messina Denaro e Michele Zagaria, non credo che passeranno un Natale tranquillo e felice, visti i recenti, brillanti risultati delle forze dell'ordine). Forze dell'ordine che svolgono brillantemente il loro lavoro, alle quali vanno i sinceri e meritati complimenti della Lega Nord, soprattutto in un periodo particolare come quello che stiamo vivendo di effervescenza sociale, spesso strumentalizzata anche politicamente, bisogna riconoscerlo. Gli elogi vanno alla nostra polizia, ai nostri carabinieri, a tutte le forze dell'ordine per la loro professionalità, per la fermezza e la pacatezza dimostrate. I nostri complimenti se li meritano pienamente e, visto il periodo particolare, anche gli auguri di buon Natale. In questo scenario, il provvedimento che stiamo per approvare porterà sicuramente ulteriori benefici nella lotta alla criminalità. Una criminalità in evoluzione, che si sta modernizzando e che è sempre più da difficile da affrontare e sconfiggere

In questo difficile percorso di lotta e di contrasto alla criminalità, noi della Lega Nord siamo convinti ci sia bisogno dell'apporto e della condivisione di tutte le forze politiche;

In questo ragionamento, è doverosa una riflessione sui tanti benefici cui può portare una seria lotta alla criminalità e alla mafia: benefici sicuri per il nostro Paese,

A noi della Lega Nord piace pensare ad un Sud libero dalla criminalità organizzata e dalle organizzazioni mafiose, ad un Sud che attira investimenti, che rilancia la propria economia, che sviluppa il suo territorio nel campo del turismo, ad un Sud che rispetta e valorizza il suo straordinario patrimonio ambientale, così come voleva fare il sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, un esempio per tutti gli amministratori del nostro Paese. Angelo Vassallo voleva la lotta alla mafia e una buona amministrazione, perché al nostro Paese servono la lotta alla mafia, la responsabilizzazione degli amministratori amministratori e il federalismo fiscale, quello che vuole da sempre il nostro movimento, la Lega Nord. Solo così rilanceremo l'economia e l'occupazione nel Sud del nostro Paese; solo così permetteremo agli investitori economici di impegnare risorse anche nel Meridione;

Una delle eccellenze realizzate dal ministro dell'interno Maroni è sicuramente l'Agenzia per la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla mafia: è giusto e doveroso ricordarlo. Basti pensare ai numeri che sta ottenendo: oltre 18 miliardi di beni sequestrati e confiscati. C'è voluto un Ministro come Maroni, c'è voluto questo Governo per realizzare quell'Agenzia, che era - ricordiamocelo - il sogno di gente come gli indimenticati Pio La Torre, come il generale Dalla Chiesa, i giudici Falcone e Borsellino. Credo che oggi il miglior modo per onorare la memoria di queste persone sia quello di poter elencare, sequestro dopo sequestro, i tanti beni sottratti alle cosche mafiose. Questa è la filosofia della Lega Nord, che preferisce gli Nord, che preferisce gli arresti e i successi della squadra catturandi ai tanti convegni sulla mafia che vengono fatti in questo Paese, che preferisce ascoltare l'elenco

per noi, la frase «Vieni via con me» ricorda una data, quel mercoledì 17 novembre di quest'anno, in quel di Casal di Principe, quando un agente della famosa squadra catturandi, dopo aver ammanettato il pericolosissimo e supermafioso Antonio Iovine, gli disse: «Uè

disorganiche e delle carenze sulle quali bisogna riflettere. Bisogna però anche cogliere l'occasione per esaltare il momento collaborativo emblematicamente assunto dai partiti dell'opposizione, e quindi in particolare dal Partito Democratico, con il ritiro di tutti gli emendamenti sulla base di un accordo raggiunto sin dal recepimento dell'ordine del giorno del 3 agosto scorso, in occasione della approvazione, peraltro all'unanimità, del disegno di legge relativo al cosiddetto codice antimafia, anche in quell'occasione, grazie ad un coerente contributo di idee e di esperienze del Partito Democratico. Quell'ordine del giorno, sottoscritto da tutti i Gruppi parlamentari e recepito dal Governo, costituisce oggi la base per un rinnovato impegno e per un'intensa attività parlamentare per consentire di aggiungere in tempi rapidi, in verità molto rapidi, un ulteriore tassello alla manovra d'aggiornamento. Il dibattito su questo disegno di legge avvenuto nella giornata di ieri ha conosciuto momenti di forte tensione forse un momento di riflessione e autocritica da parte di tutti, signora Presidente e onorevoli colleghi, sia necessario per auspicare un rinnovato clima di confronto su una tematica quanto mai complessa come questa in trattazione e che sta a cuore a tutto il Parlamento. Non si può non dare atto atto alla nostra Capogruppo, la senatrice Finocchiaro, al presidente Vizzini e al Ministro dell'interno, che peraltro è intervenuto tempestivamente questa mattina nella seduta

I 10 articoli, nonostante la caratteristica di disorganicità del decreto-legge in esame, e lo stesso ordine del giorno del 3 agosto offrono notevolissimi spunti per il lavoro che attende le due Commissioni competenti e sollecitano il recupero di numerosi disegni di legge già presentati dalla maggioranza, dal Partito Democratico e dagli altri partiti di opposizione. È inutile qui ricordarli: sarà compito poi del Comitato ristretto selezionarli, individuarli e renderli coerenti con la grande strategia di contrasto alle mafie attraverso il disegno di legge recentemente presentato dal Governo. È forse questa un'occasione irripetibile per intervenire anche su quella prevenzione generalista che necessariamente deve accompagnare la straordinaria azione di repressione di repressione della magistratura e degli organismi investigativi delle forze di polizia e che esige la lungimiranza della politica e della pubblica amministrazione. un'occasione irripetibile anche per dare organicità alla produzione, all'aggiornamento, alla raccolta delle norme del settore, chiudendo definitivamente la stagione della frenetica, emergenziale e disorganica attività legislativa. In questo, il Partito Democratico darà ancora una volta prova di quella sensibilità sul tema della sicurezza che ha sempre caratterizzato la sua azione politica, esaltando la professionalità, la dignità e l'abnegazione di tutte le donne e di tutti gli uomini delle forze di polizia. A loro, signora Presidente, onorevoli colleghi, va tutta la mia ammirazione e il mio rispetto.

che andremo ad arricchire nei modi che abbiamo concordato: in quell'occasione, infatti, riprenderemo questo lavoro e lo porteremo avanti su altri fronti. Il dato che ritengo estremamente positivo, come accennava il senatore De Sena, è che si sia riusciti a lavorare bene insieme, pur in ore tempestose

Vorrei dire che non ci sono stati i soliti voli di falchi e di colombe che da qualche mese portano il nostro vivere alla esasperazione ornitologica. Siamo riusciti a vedere con simpatia, ragionando, un decreto-legge del Governo.

vede l'immediato intervento su norme di recente fattura. Credo che il Parlamento abbia il dovere di intervenire per migliorare e interpretare le norme approvate uno, due o tre mesi dopo

di una commissione ministeriale per l'individuazione dei punti da riformare del codice di procedura penale del 1989, ricordo che mettemmo insieme un meccanismo che imponeva ai magistrati, vi fosse un contrasto di giurisprudenza a qualsiasi livello (a iniziare dai pretori), di informare il Parlamento affinché intervenisse. La norma era talmente di buon senso che ovviamente fu lasciata in un cassetto, e non se ne parlò più.

dal ministro Maroni, dai suoi Sottosegretari, dal Sottosegretario alla giustizia e da tutti coloro che ci hanno messo impegno e cuore, perché siamo tutti d'accordo nel contrastare la criminalità. Siamo partiti da un provvedimento, il primo decreto sicurezza, abbiamo affiancato la legge sulla sicurezza. Non sono stati momenti da poco. Abbiamo lavorato tanto, abbiamo condiviso determinate problematiche con l'opposizione

abbiamo discusso a lungo sulla norma che penalizza i comportamenti degli imprenditori quando non denunciano le pressioni di stampo mafioso.

Alla fine però, proprio per rendere più efficace la lotta alla mafia, abbiamo approvato quella norma. E così via. Non c'è dubbio che martedì inizieremo a discutere il provvedimento nel quale

non avranno luogo, e la giornata sarà riservata ai lavori delle Commissioni, con particolare riguardo ai provvedimenti previsti dal calendario per la prossima settimana. Come già comunicato, Come già comunicato, l'Assemblea tornerà a riunirsi venerdì 17 dicembre, alle ore 11,30, per l'informativa del Ministro dell'interno sugli incidenti avvenuti a Roma nella giornata di ieri.

Grazie